Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto magistrale statale «Guido Dorso» di Ariano Irpino, in Provincia di Avellino ai quali rivolgiamo il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio.

Al fine di procedere con maggiore chiarezza, chiedo due cose: ai colleghi del Senato silenzio e attenzione ed al relatore e alla rappresentante del Governo di esprimere nuovamente il proprio parere sugli emendamenti

ha detto, era stato accantonato l'articolo 32. Poiché le ragioni che hanno determinato

sul quale era stata richiesta una riflessione ulteriore, le chiedo di poter ricominciare dall'articolo 32 per poi esprimere il parere sugli

dal seguente*: "Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello il cui numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti fra gli iscritti ad un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto"». comma risulta così formulata: «In tutti i distretti il voto è comunque espresso per un solo candidato. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica».

«il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché presso gli uffici giudiziari, deve essere svolto a titolo gratuito». Quindi è evidente che, quando è condizionato ad una riformulazione,

l'articolo 39, che rappresenta un punto certamente rilevante della riforma; parliamo delle modalità di svolgimento del tirocinio. Nell'articolo 39 è prevista innanzitutto una preselezione. Riteniamo che questo sia un istituto da evitare perché inutile e dannoso; dannoso rispetto ad una selezione che non può che colpire quella fascia giovanile di laureati che partono già in condizione di svantaggio sociale di svantaggio sociale e economico, di preparazione nel complesso. Abbiamo dei laureati che aspirano ad entrare nella professione legale. Ebbene, si regola con legge il modo con cui si svolge il tirocinio; non si comprende la necessità di una selezione preventiva con strumenti informatici, con testi non meglio identificati, che mira certamente a tagliare e ad escludere - io direi

soggetti non per ragioni attinenti alla selezione qualitativa, alla selezione diretta a stabilire la presenza di preparazione, di tendenze e di attitudini. Siamo quindi a strumenti che io definisco trancianti, strumenti che in maniera piuttosto superficiale e arbitraria, dannosa quindi, ingiusta più che altro, escludono soggetti che potrebbero essere alla prova dei fatti anche migliori di quelli cui viene consentito di proseguire oltre. Non crediamo quindi che questa preselezione possa servire all'obiettivo che è comune: quello di migliorare la professione forense, di incidere anche sul numero eccezionalmente alto di avvocati che abbiamo nel nostro Paese. Ma questa riduzione del numero non può essere fatta in maniera arbitraria, in maniera sbagliata, in modo ingiusto e così preliminare. Dobbiamo consentire a tutti, come vuole la nostra Costituzione, l'accesso alla professione, e la selezione deve essere basata su prove che scaturiscano da un esercizio effettivo del tirocinio, che intervengano quando l'attività di preparazione si è compiuta, quando il giovane aspirante a questa professione dimostri di aver acquisito quel livello culturale che si richiede, che è preteso, e quando dimostri tutte le altre qualità che noi ci auguriamo vengano individuate, valutate e accertate in esito al tirocinio. Quindi siamo decisamente contrari alla prova selettiva.

essenzialmente, se non esclusivamente, ad un addestramento tecnico e giuridico, tralasciando un aspetto qualitativo che noi poniamo in evidenza nel comma 1 dell'articolo 39 proposto nel nostro emendamento. avvocato è «finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare principi etici e regole deontologiche». Credo che tale previsione sia un sostanziale

rappresenti un elemento maggiormente qualificante per la stessa professione, per lo stesso Consiglio nazionale forense, che non può essere lasciato arbitro. A mio giudizio, la posizione che l'articolo riconosce al Consiglio quale assoluto vertice ed esclusivo organismo competente a regolare tutta l'attività del tirocinio, che rappresenta una parte

restringere i confini della propria organizzazione e della propria struttura limitando i confini tutti all'interno. Vorrei sottolineare un

presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte d'appello. A proposito di quest'ultimo punto, penso a quanto potrebbe essere utile il tirocinio sviluppato anche presso il famoso, agognato ufficio per il processo, previsto in alcuni nostri progetti di legge e che mi auguro che un prossimo Governo, più sensibile alla riforma della giustizia, possa al più presto varare. limitiamo a due i praticanti che possono esercitare l'attività di tirocinio presso uno studio legale. Intendiamo quindi contribuire a una svolta che dovrebbe essere di grande qualità: superare la pletora di praticanti che oggi affollano i grandi studi professionali, con la conseguenza di un sostanziale e pratico abbandono di tutti questi giovani a se stessi, salvo rare eccezioni la cui valutazione lascio immaginare di solito su cosa sia fondata.

noi teniamo a sottolineare che giustamente viene abolita la prova di preselezione per l'accesso alla pratica, ma vi è stata una lunga e laboriosa fatica per arrivare a questo punto e siamo lietissimi che finalmente la maggioranza abbia recepito questa proposta. *(Applausi del senatore Perduca intervento sull'emendamento 39.200 che avevamo manifestato questa volontà fin dell'inizio per impedire che ai giovani fosse vietato l'accesso alla professione legale attraverso una prova preselettiva irragionevole. Quindi, voteremo chiaramente con la Commissione, però

sul suo contenuto e sul suo carattere straordinariamente discriminatorio rispetto a categorie di soggetti che legittimamente potrebbero voler intraprendere la professione legale: «Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previste per l'avvocato dagli articoli 17 e 18». In definitiva, stando a questo comma, il giovane - o anche il non giovane o giovanissimo - che intenda o desideri dedicarsi alla professione di avvocato deve tagliare i ponti con qualsiasi attività diversa da un lavoro subordinato di tipo privato. Prescindo da ogni considerazione, che pur potrei fare sull'inspiegabilità della discriminazione (sarebbe molto interessante sentire una convincente spiegazione

Chi lavora in un'amministrazione pubblica, chi fa il professore, il funzionario, o anche soltanto chi svolge funzioni che un tempo si chiamavano di concetto, si vede completamente preclusa la possibilità di entrare in un percorso che ipoteticamente potrebbe portarlo, in seguito, all'esercizio della professione legale. Credo che ciò sia veramente ingiusto, incomprensibile e sostanzialmente inaccettabile ed è per questo motivo che abbiamo proposto l'emendamento, in favore del quale voteremo convinti. La richiesta di voto elettronico è già

la condizione di affrancamento del giovane che svolge il tirocinio da un'occupazione che possa distoglierlo, non si riesce a capire per qual motivo il lavoro privato è compatibile con il tirocinio e il lavoro pubblico, che può anche essere a tempo parziale o con contratti precari, dovrebbe essere invece incompatibile. Ritengo che l'articolo 39, al comma 8, preveda già il controllo dell'effettività del tirocinio,

nella seduta antimeridiana, dopo i voti sulle risoluzioni riferite al progetto di Programma nazionale di riforma, il senatore Azzollini ha proposto una serie di riformulazioni alla mozione n. 314 dei senatori Rutelli ed altri. Al fine di consentire una più agevole lettura dei testi da parte dell'Assemblea, le predette proposte di modifica sono state riportate in un testo a fronte che è stato distribuito.

A questo punto, chiederei al senatore Rutelli se accetta le riformulazioni alla sua mozione proposte dal senatore Azzollini, con l'intesa che le proposte di modifica che lei non dovesse accogliere, ove mantenute dal senatore Azzollini,

nel corso della discussione precedente, salvo ve ne sia la necessità per interventi politici da parte dei colleghi.

Presidente, ringrazio il presidente Rutelli, perché mi pare che sostanzialmente accolga l'insieme delle riformulazioni che gli avevo proposto. Penso che egli abbia intenzione di

dove egli chiede l'istituzione di una commissione composta da personalità per un parere *pro veritate* sulla questione dell'energia nucleare. Su quest'ultimo, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà in Signor Presidente, volevo solo comunicare i motivi per i quali non parteciperò al voto, in dissenso dal mio Gruppo, su questa mozione, che considero, più che una mozione, un programma di Governo del collega Rutelli. Semplicemente, in quanto senatore eletto per la circocoscrizione Estero, io non posso non tener conto del fatto che una delle prime azioni del nuovo partito politico del senatore Rutelli alla Camera è stata, il 23 giugno di quest'anno, la presentazione di un disegno di legge per la soppressione della circoscrizione Estero.

reintrodotto contro l'esito del *referendum* del 1993. Credo che iniziare a chiamare le cose con il loro nome possa sicuramente andare nella direzione di promuovere delle radicali riforme, che purtroppo

Immagino che la mozione dovesse avere un senso complessivo e una struttura logica, invece ne vengono smembrate parti. Non sappiamo quale tipo di impianto andiamo a votare. Mi sento estremamente sconcertato, e credo che sia sconcertata la maggioranza dei colleghi in questa Aula. Stiamo votando qualcosa di cui non sappiamo quale sarà l'insieme.

a deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento per motivare il proprio orientamento. Tutto è rispettabile; osservo soltanto che qui c'è un testo scritto, che può essere condiviso per alcune parti, meno per altre, dire, è stampato e distribuito ed è caratterizzato da alcune limitate differenze rispetto al testo originario. Lo dico molto tranquillamente al collega Livi Bacci: se lui dovesse adottare questo criterio con tanta solennità a proposito del provvedimento sull'avvocatura che stiamo votando, e che lui continuerà a votare tra cinque minuti, ci sarebbe da ridere. È la terza volta che l'Aula del Senato discute questa mozione; è disponibile un testo da settimane.

consideri questo testo come se non esistesse più: esiste, è solido, è importante; ci possono essere punti di dissenso, come quello annunciato adesso dal collega Legnini, ma pregherei di non dipingerlo per quello che non è. Ha una sua coerenza e un suo significato; ovviamente lo si può non condividere, ma non affermando che non c'è. C'è, è modificato per alcune parti e, come si suol dire nel lessico parlamentare, stampato, distribuito, leggibile e votabile: chi non lo vuol votare francamente trovi un argomento di merito e non quello puramente formalistico che ho appena sentito. *(Applausi

L'argomento del senatore Livi Bacci è assolutamente non comprensibile, a meno che non si voglia applicare questo suo sconcerto, come già stato anticipato, per la verità in sintesi, dal senatore Rutelli, a tutte le attività che svolgiamo in questa Aula quando dobbiamo votare emendamenti ad un articolo oppure articoli della stessa legge. [DE

a nostro avviso va invece mantenuto perché dà un'indicazione finalmente concreta sul tema delle liberalizzazioni nel nostro Paese. Oltretutto è rispondente non ad una parte politica ma all'indicazione istituzionale dell'*Antitrust*.

più ampie liberalizzazioni nel nostro Paese.

e quali investimenti effettivamente si metteranno in moto. La richiesta è che il Governo indichi, in questo momento di grave crisi economica e di scarsità di mezzi, le priorità sulle quali concentrare le politiche delle opere pubbliche, pubbliche, piccole, medie e grandi. Mi pare una proposta sinceramente condivisibile, che sarebbe ben accolta da tutti i settori interessati, oltre che dagli enti territoriali.

Governo ad esprimersi, mira alla soppressione della lettera *o)*, che recita: «va istituita un commissione composta da 10 personalità indipendenti (economisti, tecnologi, scienziati) che entro quattro mesi metta a disposizione del Parlamento un parere *pro veritate* sulla fattibilità economica e tecnologica della proposta del nuovo nucleare italiano».

39.901/2, 39.901/3, 39.901/4,

un sussulto di dignità in difesa delle nostre comuni prerogative. Noi siamo qui a discutere, ma io vorrei leggere molto rapidamente

che ci fa sapere che questo Governo, che lui rappresenta *pro tempore*, in queste ultime ore ha prospettive di tempo che sembrano restringersi non ad anni

dell'attuazione del programma Rotondi, che considera conclusa la nostra legislatura e ci annuncia che ormai non ci sono più le condizioni per andare avanti. le chiedo formalmente di far venire in Senato questi signori e il Presidente del Consiglio per mettere ordine e fare chiarezza su tali aspetti.

ha chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio. Questo per noi apre un *vulnus* istituzionale e costituzionale. *(IdV)*. Faremo un corso di formazione a chi non sa parlare e pensa solo ad ululare. Siamo pronti a dare un po' di spiegazioni. Dopodiché... scoperto, è un nervo scoperto, perché è il fallimento di una coalizione che deve andare a casa!

Presidente, la verifica del numero legale è una procedura che consente all'opposizione di effettuare una sua funzione. a questa verifica corrisponde un'alterazione dei voti, come visibilmente si vede, lei ci deve dire cosa dobbiamo fare: dire i nomi dei senatori che non ci sono, chiedere ai Segretari di scendere dal banco della Presidenza? Ma se i Segretari autonomamente decidono di non farlo, noi da chi siamo tutelati? A chi dobbiamo chiederlo? *(Applausi

che è impossibile per i senatori Segretari provvedere alla verifica dei senatori presenti se la votazione è chiusa. Non abbiamo avuto il tempo in questa occasione ...

PRESIDENTE. La prima verifica del numero legale l'ho dichiarata chiusa e il Senato era in numero legale. Non posso verificarla nuovamente

... LEGNINI *(PD)*. No. Forse non mi sono spiegato: c'è una disposizione in questo senso. Noi stiamo per votare; prima di votare, numero legale o voto elettronico, poco importa, si assicuri che

Ovviamente lo faccio al momento del voto. *(Proteste del senatore Ferrara)*. Senatore Ferrara, siccome prima mi è stato detto che non si poteva perché avevo fatto troppo in fretta, vediamo di andare per ordine.

si presuppone che il collega sia in Aula o nei pressi avendo inserito la scheda. Eventualmente il controllo si può fare nel momento in cui si vota

Grazie

si possa svolgere nello studio di un avvocato che abbia un'anzianità di almeno due anni. Ciò sarebbe ancor più importante perché

potrebbe apparire un dettaglio: la norma di cui ci siamo occupando prevede infatti la possibilità di un tirocinio, per chi voglia diventare avvocato, presso un ufficio giudiziario, ma si scopre che, inopinatamente, questo tirocinio non può durare più di dodici mesi. Perché questa previsione? Esiste una ragione che abbia a che fare con la qualità della formazione che un ufficio giudiziario può dare a un giovane nella prospettiva che egli, o ella, diventi avvocato? Direi di no, perché è negli uffici giudiziari che confluisce l'attività dell'avvocato e direi che il tirocinio presso un ufficio giudiziario offre uno spettro di esperienze e di opportunità professionali

sapore più o meno velatamente ideologico, perché essa allude a un'incomprensibile diffidenza e a un principio di contrapposizione fra l'ambito della professione legale e l'ambito delle attività che si svolgono negli uffici giudiziari, che crediamo sia da respingere, come fatto culturale prima ancora che come scelta tecnica. Chiediamo quindi un "sì" su questo emendamento e ne chiediamo altresì

il tenere fermo un limite di dodici mesi obbedisce ad una logica. Poiché la possibilità di tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato e gli uffici giudiziari

blocchiamo la possibilità di tirocinio per migliaia di giovani. Noi dobbiamo aiutare i giovani a svolgere il tirocinio; quindi il termine di dodici mesi ha una sua logica. LONGO *(PdL)*. Signore e signori del Senato, io credo che vi sia una diffusa mancanza di informazione sulla formazione dei giovani avvocati.

certamente i più intelligenti; ammettiamolo pure. Ma la formazione del giovane avvocato comincia così: «Intanto, caro, vieni con me, che ti mostro dove son tutte le cancellerie. Poi partecipi agli incontri con i clienti che arrivano e ti dicono che vogliono denunciare il vicino di casa perché non li ha salutati». La formazione, quindi, non è una formazione soltanto tecnico‑giuridica; è la formazione artigianale che fa dell'avvocato un grande artigiano e del grande avvocato un grande artista. Non si può fare una formazione di andando negli uffici giudiziari, senza sapere cos'è il vero e proprio contatto con il pubblico, che gli uffici giudiziari - ahimè - non hanno, o hanno con caratteristiche completamente diverse da quelle, umanissime, del contatto diretto che ha l'avvocato.

Il nostro emendamento mira a rimuovere il limite temporale per la pratica svolta presso sedi estere (uffici dell'Unione europea o studi legali all'estero). Anche in questo caso, ci poniamo nella prospettiva di una professione legale lanciata verso il futuro piuttosto che ripiegata verso il passato del piccolo e a volte polveroso studio professionale, in cui qualche volta si impara un buon artigianato e qualche volta si è invece circoscritti in una dimensione non ariosa della professione del giurista e dell'avvocato come ci piace pensarlo, cioè come un professionista capace di offrire un servizio ai cittadini e capace di collocarsi sull'onda delle trasformazioni della società. Ebbene, in questa prospettiva, che è la nostra e che, rispettabilmente, si può non condividere, nella consapevolezza che c'è qualcosa che appartiene al passato e qualcosa che appartiene al futuro (e queste norme certamente al futuro non appartengono), noi chiediamo di votare «si» su questo emendamento

l'emendamento è ammissibile aggiungendo, come chiede la Commissione bilancio, la seguente frase: «Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici,

Signora Presidente, siccome abbiamo sentito evocare non soltanto i giovani ma anche le botteghe artigiane, con la speranza che arrivino, addirittura, a produrre degli artisti, si ritiene che quante più botteghe artigiane si possono frequentare, tanto più l'arte potrà essere, in effetti, composta. Si è proibito un soggiorno all'estero superiore ai sei mesi. Speriamo, invece, che le nostre botteghe

a richiesta del praticante e su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso in cui si possa presumere che la mole di lavoro di uno dei due non sia tale da permettere al praticante una sufficiente

Grazie favorevole del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento che riguarda i giovani avvocati. L'emendamento semplicemente fa riferimento ai praticanti avvocati e alla necessità che, oltre al rimborso delle spese, venga dato un compenso adeguato e commisurato all'apporto dato per l'attività svolta. Crediamo che questa sia una proposta di equità e di giustizia e, quindi, chiediamo che, pur accettando la formulazione

perché, in effetti, il problema, posto poc'anzi anche dal senatore Casson, deve essere ricordato. Da una parte si ricorda l'importanza e la nobiltà della professione forense rievocando anche i rilievi costituzionali, dall'altra la si vuole trattare come l'artigianato. anche l'artigianato avrà bisogno delle sue misure relative al tirocinio, i senatori Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva e Villari chiedono che il tirocinio professionale non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale il titolare dello studio legale riconosca al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito dell'attività di tirocinio. È vero che più avanti voteremo un emendamento della Commissione in cui si parlerà di un rimborso forfetario, pur se a partire dal secondo anno, si sa però, in virtù delle difficoltà dell'inizio del tirocinio ricordate poco fa dal senatore Longo, che comunque la mole di lavoro è tale anche dopo i primi mesi quando si è fatto

che l'emendamento prevede che «al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio». Questo era evidente, non occorreva scriverlo, ma la Commissione lo ha scritto. È soltanto il riconoscimento di un rimborso commisurato all'attività svolta per conto dello studio, che nasce necessariamente dal secondo anno

le posso rileggere il parere. ICHINO *(PD)*. Ho capito, ma qui non c'è nessuna implicazione rilevante sul piano finanziario. PRESIDENTE. Io però non posso personalmente contestare l'espressione di una Commissione.

*(PD)*. Questo emendamento dice soltanto che la preclusione della qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato è la regola: l'espressione "di norma" significa che, se le cose si svolgono regolarmente, il rapporto non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato. Sappiamo che, accade diffusamente che invece si verifichino degli abusi; per esempio, che lo studio legale poco serio utilizzi il giovane, sotto la forma di un rapporto di praticantato, in realtà facendogli fare

ovviamente non può mettere in discussione il parere della Commissione bilancio, che le leggo: «In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte

se questo accade, il dirigente responsabile risponderà del danno erariale prodotto; ma non è consentito escludere che chi è vittima di questa simulazione fraudolenta possa agire in giudizio per il suo riconoscimento.

questo emendamento determinerebbe una sovraesposizione finanziaria per il bilancio dello Stato.

distinguendo la pratica forense, e quindi queste forme di collaborazione che non determinano un rapporto di lavoro subordinato, dalla simulazione di rapporti di pratica e collaborazione, che invece sono una forma di sfruttamento dei giovani avvocati. Credo che questo sia un modo equilibrato per

che il suo ragionamento potrebbe essere valido soltanto se l'argomento riguardasse l'instaurazione di rapporti di lavoro all'interno di studi prettamente privati. *(Il senatore D'Alia è al telefono)*. Però se il presidente D'Alia non mi ascolta è inutile che io intervenga.

consentirà agli oratori di intervenire anche oltre i cinque minuti stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, cercando comunque di armonizzare i tempi nel rispetto dell'orario previsto per la chiusura della seduta.

gravi vicende che hanno interessato diverse Regioni del nostro Paese nel corso della prima settimana del mese di novembre. Vorrei cogliere l'occasione per fornire anche alcune informazioni in merito alla situazione di maltempo

comuni come Angri, San Marzano sul Sarno, Nocera inferiore, Nocera superiore, Capaccio, San Pietro al Tanagro, Sala Consilina, Santa Cecilia di Eboli. Numerose sono state le esondazioni, soprattutto di fiumi e torrenti del reticolo idrografico minore. In particolare si è registrata una situazione critica per quanto riguarda il fiume Sele, che in molte zone è esondato, determinando gravi difficoltà per l'acquedotto del Sele, che fornisce, com'è noto, acqua a tutto il comune di Salerno e ad altri numerosi comuni circostanti. Allo stato attuale, si sta organizzando un sistema di approvvigionamento idrico alternativo. In base alle informazioni che abbiamo ricevuto, a causa dei danni che l'acquedotto ha subìto, saranno necessari interventi per diversi giorni, forse per alcune settimane che, se si lavorerà ventiquattr'ore al giorno, potranno ripristinare la fornitura di acqua potabile nell'arco dei prossimi 15 o 20 giorni. Al momento, sono 500.000

cautelativo, dai numerosi comuni che ho citato, per evitare che la situazione potesse degenerare. Stiamo seguendo e monitorando la vicenda. La protezione civile della regione e ovviamente i Vigili del fuoco e tutte le altre strutture del sistema nazionale di protezione civile sono sul posto per cercare di fronteggiare anche questa ennesima situazione di difficoltà. Per quanto riguarda, invece, le vicende meteorologiche che hanno interessato agli inizi del mese numerose regioni italiane, sappiamo purtroppo che sei sono le persone che hanno perso la vita a causa di quello che è accaduto: due sono morte nel vicentino, tre nel comune di Massa, una a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, mentre c'è ancora un disperso a Rovigo. Il maltempo ha determinato l'allontanamento di migliaia di persone, gravi danni con alluvioni, smottamenti, frane, interruzione alla viabilità provinciale e comunale, ma anche nazionale, se si pensa alla vicenda dell'autostrada Milano-Venezia, che è rimasta chiusa al traffico nel tratto Montebello-Soave praticamente per tre giorni. Le province maggiormente interessate sono state quelle di Milano, Brescia, Mantova;

Cosa è stato fatto preventivamente, e poi durante l'emergenza? Il Dipartimento già il 30 e il 31 ottobre aveva emanato i vari avvisi di condizioni meteorologiche avverse, dando segnali di forte criticità di precipitazioni nelle regioni che ho citato e poi di grave rischio idrogeologico, in particolare in Friuli, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise.

e poi nel corso della giornata tutta la regione Veneto, comprese quindi anche le province di Padova, di Treviso e di Belluno. Sulla base di questi avvisi, le varie Regioni si sono organizzate per cercare di fronteggiare le possibili situazioni di crisi. Ricordo che ogni Regione che ho citato è dotata di una sua struttura di monitoraggio e di previsione meteorologica ed è autonoma nell'emissione successiva agli avvisi nazionali per quello che riguarda il territorio circostante. La Regione Veneto emanava, in conseguenza di queste previsioni meteorologiche, anche i propri avvisi di criticità, trasmettendoli a prefetture e Comuni interessati. I primi momenti, la notte fra il 31 ottobre e il 1° novembre, com'è noto, le situazioni più critiche hanno riguardato la Toscana, dove purtroppo, nella provincia di Massa, per una colata di fango e di detriti una casa è stata travolta e tre persone hanno perso la vita. L'attenzione si è concentrata in quel momento soprattutto in quell'area per l'organizzazione dei soccorsi e anche per quello che riguarda l'attenzione dei *mass media* che hanno dato ampio risalto alla vicenda di Massa, così come hanno dato risalto all'interruzione ferroviaria che aveva riguardato in Liguria il tratto ferroviario fra Ventimiglia e Savona. e Savona. Nello stesso tempo cominciava già ad emergere la criticità che riguardava il Veneto, in particolare per quello che all'inizio interessava la provincia di Verona, con il Tramigna che esondava a a Soave e l'Alpone che cominciava a creare una serie di difficoltà nelle località circostanti. Anche il Bacchiglione raggiungeva il livello di guardia a Vicenza e si poteva considerare il rischio che pure il Livenza, al confine fra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, potesse arrivare a dei livelli che non erano stati riscontrati negli ultimi Le piene che hanno riguardato il Bacchiglione e il Livenza in particolare sono ultracentennali, come si usa dire, e quindi l'evento che abbiamo dovuto fronteggiare è stato di carattere assolutamente eccezionale. A livello locale si sono organizzate le attività di monitoraggio e soccorso inizialmente nella provincia di Verona, dove nell'ambito della prefettura sono stati costituiti i centri di coordinamento e soccorso. Lo stesso è successo a Vicenza,

i sindaci dei Comuni interessati e il presidente della Provincia e si cominciavano a coordinare le attività di soccorso. La sera del 1° novembre la situazione veniva riferita dalle autorità locali come sotto controllo nella provincia di Verona e di Vicenza e non si registravano ancora situazioni particolarmente critiche in quella di Padova. Io stesso mi sono messo in contatto la sera del 1° novembre con il sindaco di Vicenza, il sindaco di Padova, le varie autorità prefettizie delle tre Province. Avendo riscontrato che le informazioni che ricevevamo non corrispondevano a quelle che mi venivano date in tempo reale dai personaggi e dalle istituzioni con le cui mi ero messo in contatto, attivavo tutta una serie di iniziative finalizzate a far convergere in queste tre province una serie di squadre, di colonne mobili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e in particolare anche delle Forze armate, con il Genio militare, che convergeva da tre Regioni limitrofe, inviando immediatamente a Vicenza, nel corso alla stessa notte, oltre 150 unità unità dotate di mezzi anfibi, idrovore e mezzi necessari alla gestione di questa emergenza. la provincia di Massa, con la Liguria, nonché con la Calabria e il Friuli-Venezia Giulia, ossia le regioni che nel frattempo venivano interessate da un'ondata di maltempo.

Mi sono poi trasferito nella provincia di Verona. Sono stato a Monteforte d'Alpone per verificare direttamente la situazione, che mi era stata descritta come una delle più critiche.

a seguito di una legge regionale (visto che la protezione civile è materia di legislazione concorrente), la gestione della materia della protezione civile è stata affidata direttamente alle Province, che devono avere la responsabilità, il ruolo e il compito di fungere da punto di coordinamento per tutte le problematiche in tale ambito. Siccome la situazione era particolarmente critica, sebbene non richiesto, ho lasciato nelle tre

2 novembre, si creassero delle situazioni estremamente critiche anche per la viabilità ed il trasporto. Grazie al lavoro della Polizia stradale, delle società competenti e di tutte le organizzazioni di volontariato e delle polizie municipali e locali, vi è stata una gestione mirabile della situazione legata al traffico. A Verona, oltretutto, nei giorni immediatamente successivi, doveva svolgersi la più importante fiera europea

lo stesso accadeva anche a Monteforte d'Alpone, a Soave. San Bonifacio era stata molto meno coinvolta. A Cresole, dove si è purtroppo registrata una vittima, la situazione era un po' più complicata, perché il Bacchiglione aveva rotto gli argini in due punti strategici e quindi l'intervento di rimozione dell'acqua e del fango è stato più lento, ma efficace.

nazionale, i Vigili del fuoco hanno partecipato inviando colonne mobili dal Piemonte, dal Friuli, dalla Lombardia, dall'Emilia-Romagna, dalla Liguria; ma anche dalle Marche, dall'Abruzzo, dalla Toscana sono partiti mezzi di movimento terra, mezzi nautici e anfibi. Lo stesso vale per le Forze armate, che hanno hanno rappresentato una organizzazione davvero efficace, inviando oltre 250 unità con 28 mezzi dalle province di Verona, di Vicenza e di Padova. Nel corso dei giorni successivi c'è stato anche un incremento della presenza delle Forze armate man mano pervenivano anche sul posto, sempre coordinate e convocate dal Dipartimento nazionale su richiesta della Regione Veneto, le colonne mobili regionali; come sapete, anche a livello regionale c'è un'organizzazione che prevede l'impiego di personale di volontariato in grado di prestare assistenza in ordine alle situazioni di maggiore crisi. Le prime a intervenire sono state la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia; si sono aggiunte successivamente l'Emilia-Romagna, la Provincia Autonoma di Trento, le Marche, il Piemonte, la Lombardia. Sono arrivati complessivamente circa 250 tra funzionari e volontari, con pompe idrovore, torri faro, mezzi per la pulizia delle strade.

è la misura del territorio che ha riguardato la Bassa padovana, che è stata maggiormente colpita, come dicevo, nel comune di Bovolenta. veniva gestita e messa sotto controllo da parte delle autorità locali, si è provveduto a recuperare e a risolvere il problema degli allagamenti. Ci saranno state sicuramente delle situazioni di di difficoltà a livello anche individuale di fattorie o di imprese, ma comunque, quando mi sono recato per la seconda volta, per verificare l'andamento delle attività, in Veneto e ho effettuato dei sopralluoghi sia a Padova che a Verona che a Vicenza, ho potuto constatare una presenza massiccia di tutte le varie organizzazioni; ho visto un numero impressionante di idrovore in piena ho riscontrato, almeno da parte delle autorità locali (tutti i sindaci, i tre presidenti di provincia e ovviamente anche i prefetti), una generale soddisfazione per quella che è stata la modalità di intervento nell'emergenza di protezione civile. Abbiamo anche affrontato le problematiche che riguardavano la zona prealpina: vi sono state numerose frane e dissesti idrogeologici di vario genere. Soprattutto in provincia di Vicenza, nel comune di Recoaro, la frana del monte Rotolon si è riattivata e rischiava di coinvolgere oltre 200 persone della zona circostante. Anche lì abbiamo avviato un meccanismo di monitoraggio su 24 ore con personale militare e volontari. Sono arrivati poi i tecnici del CNR per riuscire a mettere sotto controllo gli eventuali spostamenti e attivare piani spedìtivi nel caso in cui dovesse essere necessaria l'evacuazione nella zona del comune di Recoaro. nella provincia di Verona sono ancora attivi i centri operativi che sono stati istituiti in prefettura e presso i comuni di Soave e di Monteforte d'Alpone. Per quanto riguarda la situazione degli sfollati in quella Provincia, sono 700 sono 700 gli abitanti che non sono ancora potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Nella provincia di Vicenza, oltre alla struttura di coordinamento della prefettura, sono attivi i centri operativi comunali di Caldogno e di Recoaro Terme. Non ci sono più problemi, come ho detto, per quanto riguarda la presenza di acqua ma comunque, nella provincia di Vicenza, sono 500 le persone che non sono ancora potute rientrare nelle proprie abitazioni. provincia di Padova, che è quella che sta uscendo con maggiore difficoltà dalla situazione di crisi, oltre alla prefettura sono attivi i centri operativi misti di Casalserugo e di Saletto che sono gestiti dalla prefettura e dalla Regione, oltre ai centri operativi comunali di Veggiano, Maserà e di San Nicolò, che sono gestiti direttamente dalle strutture comunali. Nella provincia di Padova ci sono 870 sfollati sono 870 sfollati ancora fuori casa e che hanno trovato alloggio presso amici e parenti, mentre 104 sono stati ospitati presso strutture pubbliche. Come ho detto, anche in provincia di Treviso, Rovigo e Belluno ci sono stati momenti di difficoltà, con esondazioni di torrenti, frane, dissesto idrogeologico,

agli interventi che, oltre al sopralluogo che ho fatto il 2 novembre ed il successivo fatto domenica scorsa, sono stati abbastanza tempestivi, sicuramente tempestivi per quanto riguarda l'operazione del Governo che, il 5 novembre, ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza

Come sapete, ieri c'è stata la visita del Presidente del Consiglio e del ministro Bossi, che hanno fatto sopralluoghi in tutte e tre le province e incontrato le autorità locali, accompagnati dal governatore

oggi il Presidente del Consiglio ha deliberato uno stanziamento che, in aggiunta ai 20 milioni di euro iniziali - che, ribadisco ancora, servivano solo

la stiamo trasmettendo alla Regione Veneto per l'intesa - l'ordinanza di protezione civile che è stata scritta quest'oggi con il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province interessate, la quale recita: «Primi interventi urgenti

sempre individuato nella persona del Presidente della Regione il commissario di Governo che ha il compito di stabilire nel dettaglio la stima dei danni

Ovviamente sono già previste le prime modalità di indennizzo per coloro i quali hanno subito i danni e, soprattutto, le modalità di intervento per garantire

in parallelo l'ABI ha stanziato 700 milioni di euro per garantire crediti super agevolati a tutti coloro i quali vi faranno ricorso e ha sospeso anche il pagamento dei mutui a qualsiasi titolo

le stesse ordinanze per quanto riguarda le situazioni di emergenza che hanno interessato le altre regioni che ho citato: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana

Anche per queste regioni dovranno essere individuate delle poste economiche che ovviamente non richiedono un impegno del Governo uguale a quello che abbiamo garantito per la vicenda del Veneto. È però altrettanto ovvio che, così come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, in relazione ad ogni situazione di criticità e ad ogni problema che sia stato anche creato nel corso della passata settimana in qualsiasi parte del nostro Paese, si possano garantire quelle risposte, quelle iniziative e quelle agevolazioni che diano la possibilità a tutti i vari territori che sono stati colpiti di riprendere le proprie attività nel tempo più rapido possibile. *(Applausi

a parlare il senatore Bevilacqua.

I gravi fatti di questi giorni hanno riportato alla ribalta il problema del dissesto idrogeologico. Basti pensare che nel rapporto scientifico del Consiglio nazionale dei geologi si afferma che 6 milioni di italiani vivono in zone ad elevato rischio. La Calabria ha un privilegio (in negativo, naturalmente), perché 409 Comuni su 409 sono in questa situazione di rischio idrogeologico. I fatti alluvionali degli ultimi giorni hanno interessato diverse regioni in diversi tempi: dalla Liguria, alla Toscana, al Veneto, in particolare, in questi ultimi giorni.

devastata dalle alluvioni. Vorrei innanzitutto esprimere la mia convinta solidarietà ai cittadini di quei territori colpiti dalle gravissime alluvioni degli ultimi giorni. inoltre informare il Senato - anche se lo ha già fatto il sottosegretario Bertolaso - che purtroppo anche la Regione Calabria ha dovuto avanzare richiesta, poi puntualmente accettata dal Consiglio dei ministri, per la dichiarazione da parte del Governo dello stato di emergenza, a fronte dei gravi eventi meteorologici che hanno interessato l'intero territorio regionale, in particolare nei giorni del 3 e del 4 settembre fino ai giorni La Regione Calabria, interloquendo con il Sottosegretario con delega alla Protezione civile, ha provvisoriamente quantificato i danni in oltre 300 milioni di euro. Nel ricordare quei giorni, ho in mente le immagini di intere famiglie che, in provincia di Crotone, sono riuscite a salvarsi dalla furia delle acque soltanto rifugiandosi sui tetti; di frane e smottamenti in diverse zone della provincia di Reggio Calabria; della cittadina di Gioia Tauro e dell'intera Piana, con i suoi rinomati agrumeti, inondata e devastata. Ancora, ricordo la notizia della tragica morte di un sessantenne travolto dalle acque di un torrente in piena vicino Tropea e, infine, intere cittadine della costa tirrenica devastate dalla furia delle acque. In proposito, lo scorso 28 ottobre ho depositato presso gli Uffici del Senato una mozione sottoscritta anche dai colleghi senatori Caligiuri, Valentino, Speziali, Bruno, Giordano, De Sena e Gentile - diretta ad impegnare il Governo allo stanziamento e al trasferimento alla Regione Calabria di congrue risorse per fronteggiare le numerose situazioni emergenziali che insistono

per garantire la messa in sicurezza dei territori, onde evitare il ripetersi, in futuro, di tragedie quali quelle a cui ho fatto riferimento. Concludo esprimendo la mia soddisfazione per il tempestivo sopralluogo svolto dal Presidente del Consiglio nei territori veneti colpiti. Mi auguro che con la medesima tempestività il presidente Berlusconi vorrà venire in Calabria per rendersi personalmente conto di quanto grave sia, purtroppo, la situazione anche nella mia terra. Ci aiuti il Governo a venir fuori dal fango.

signor Sottosegretario, voglio subito sgombrare il campo da un equivoco e comunque essere chiaro. Ci sono state molte polemiche sui giornali di oggi per la visita sua, del Presidente del Consiglio e del ministro Bossi, ieri, nelle zona alluvionate.

per iniziare a far fronte alle spese, ma anche per andare incontro ai cittadini, alle imprese, agli artigiani, ai commercianti e a tutti coloro che hanno subito i danni che conosciamo,

di Padova, i semplici cittadini e gli stessi sindaci (che sono stati in piedi per giorni e notti e sono stati i primi, in qualche caso, ad avvisare i cittadini di evacuare o di scappare), voglio anche dire,

più serietà. Non è vero, come si dice spesso, che siamo i più bravi nell'emergenza. Noi siamo bravissimi e siamo molto generosi nell'emergenza; ma l'emergenza deve essere un qualcosa che ci vede preparati. I piani di di allarme e le procedure di evacuazione sono piani comunali che i Comuni debbono fare da anni e che spesso non fanno. Quindi, non ci si può lamentare poi con lo Stato centrale se queste cose non vengono attuate; mi riferisco agli allarmi, ai meccanismi di avviso nelle situazioni di emergenza,

la voce. Serve lo Stato, serve la comunità nazionale, serve quell'unità, a volte vituperata, che si riscopre come valore proprio in questi momenti di difficoltà. Le promesse e gli impegni di questi giorni devono trasformarsi in fatti, altrimenti cresceranno ancora la rabbia e il rancore ipotizzando anche, da parte di qualche autorevole categoria economica (come abbiamo letto oggi), forme di protesta inutili e dannose. Lo Stato deve quindi rispondere con tempestività e vigore; il Governo può prevedere già nella legge di stabilità (oltre all'impegno di oggi) alcune forme di esenzione fiscale. È necessario comunque il massimo impegno in tutte le sedi per assicurare al Veneto tutte le risorse che merita, tenuto conto della generosità di questa Regione e del suo alto tasso di economia e di sviluppo, che va tutelato e conservato nell'interesse del sistema Paese.

e, come tale, è un Paese che ha nelle sue caratteristiche una fragilità e una vulnerabilità particolari. Se parlassi da tecnico e non da politico, direi che queste cose sono conosciute. È conosciuto il fatto che, nella gestione del territorio, nella gestione delle opere e nelle infrastrutture, tutti noi - la comunità scientifica, la comunità economica e la comunità sociale

eccezionali; perché si tratta, ancora una volta, di eventi di natura eccezionale. Tuttavia, noi possiamo evitare i moltiplicatori dei danni e dei danni e costruire un sistema, attraverso un'iniziativa politica e parlamentare, che miri sostanzialmente a prevedere un'ordinaria manutenzione della vulnerabilità del nostro territorio e una capacità di mitigare i fattori di rischio che pure si possono, in qualche modo, mitigare. Nei prossimi giorni, come Alleanza per l'Italia, noi avanzeremo una proposta in questa direzione.

mi auguro e auspico, e voterò in questo senso, in tutte le sedi in cui sarò chiamato a farlo, che la solidarietà nazionale si attivi per il Veneto: ma che si attivi concretamente.

La situazione in Calabria, e lo dico perché non vorrei che vi si trovasse il Veneto, è la seguente: ai Comuni è stato chiesto d'intervenire in emergenza; i Comuni si sono indebitati, alcuni sono a rischio fallimento, e adesso la situazione è tale che le imprese si rifiutano di intervenire in emergenza. Questo Governo è riuscito a far perdere quella credibilità indispensabile, che il sistema della protezione civile deve avere. Mi dispiace dover contraddire il Sottosegretario, ma l'attuale Governo, purtroppo, in questo settore, non ha fatto quanto ha promesso: non ha messo risorse in gioco. Io sono preoccupato perché, se dalla Calabria questo modo di procedere si estende, un Paese fragile come il nostro ha veramente di che rischiare. Io vorrei che in Veneto, in Toscana, nel Friuli, in Calabria, dove gli eventi eccezionali arrivano e dove si innesca la solidarietà nazionale, gli impegni che assume il Governo fossero realmente e concretamente rispettati.

Si è attivata immediatamente la protezione civile in provincia di Salerno, e un ringraziamento va alle forze dell'ordine, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco. Un grazie di cuore a tutti coloro i quali, in queste ore, stanno ancora lavorando.

con centinaia di milioni di colture che, purtroppo, sono andate al macero. La Coldiretti ha stimato un danno approssimativo di circa 200 milioni di danni effettivi. Oggi ho depositato un'interrogazione con la quale chiedo l'intervento del presidente Berlusconi, così come avvenuto in Veneto. Il presidente Caldoro si è immediatamente attivato con la Giunta, e in queste ore chiederà lo stato di calamità naturale. Quindi, signor Sottosegretario, noi chiediamo a lei e al presidente Berlusconi un intervento mirato: non un intervento a pioggia e non un intervento per colmare il il danno subito da qualche agricoltore. Noi le chiediamo un intervento, così come ha fatto con l'emergenza rifiuti, che risolva il problema e che non si limiti a tamponare. La provincia di Salerno sta vivendo adesso un momento particolarmente difficile, tant'è che il prefetto di Salerno ha istituito un comitato di emergenza. Si sono attivati il Presidente della Provincia, l'onorevole Cirielli, con tutta la Giunta provinciale. Noi, come salernitani e come campani, chiediamo che in questi giorni, così com'è avvenuto in Veneto, vengano immediatamente emesse le provvidenze a favore degli agricoltori,

Spero lo si faccia anche per la Basilicata e la Campania, che l'hanno chiesto. L'Italia dei Valori vuole innanzitutto esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza a tutte le famiglie che sono state colpite in questi giorni da questi eventi. modo, esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza ai giovani della protezione civile che puntualmente ogni anno in questi giorni devono intervenire per riparare ai danni per i quali questa volta non possiamo accusare

cosa fare e come intervenire. Purtroppo noi arriviamo sempre dopo. Noi abbiamo il nostro *superman* Bertolaso, il quale, a dispetto di *superman*, arriva sempre dopo: l'asteroide è già caduto quando arriva.

istituire tre commissari per il dissesto idrogeologico in Italia. Che fine hanno fatto? Che fanno? Cosa hanno fatto in questo anno? L'abbiamo votato. Fortunatamente il giorno dopo nell'Aula di Montecitorio quella stessa legge non

rispondere, dare delle risposte concrete, quando sappiamo cosa fare, dove fare e come intervenire? Non possiamo assistere puntualmente ogni anno a queste cose.

Il problema è che noi dobbiamo intervenire e arrivare prima e non possiamo farlo se non ci sono i fondi e se andiamo a sottrarre i fondi ad un Ministero, come quello dell'ambiente, che è deputato a svolgere

dottor Bertolaso (che domani lascerà), ma un'altra persona, che verrà qui a raccontarci sempre che con l'elicottero ...

non recupera il proprio ruolo di programmazione e alta direzione che l'articolo 9 della Costituzione impone a tutela del territorio, non si lamenti poi dell'accoglienza che ieri i cittadini del Veneto e dell'Abruzzo hanno riservato al Presidente del Consiglio*,* contestandolo pesantemente perché, distrutto da ben altre occupazioni e frequentazioni, sta trascurando del tutto il compito istituzionale che dovrebbe invece assolvere insieme al Governo.

in virtù della quale non ci debbono essere divisioni fra l'una o l'altra regione. Siamo tutti italiani e, purtroppo, siamo in una situazione ancora una volta di emergenza.

per quello che lei ha fatto nel tempo. Lei adesso ha fatto il Sottosegretario, si è assunto questo onere, questa responsabilità, che non è certo - almeno non l'ho intesa sinceramente come tale - una vera e propria responsabilità politica. Personalmente, ho sempre guardato a lei come ad una figura più istituzionale, che ha sempre agito per il bene del territorio.

ma credo che nessuno possa sottovalutare l'impegno che lei in questi anni ha messo nella difesa del territorio e nella valorizzazione

non possiamo certamente dirle nulla rispetto all'attività di soccorso prestata; un'attività per la quale non soltanto ringraziamo la Protezione civile, sia che si tratti della Protezione civile nazionale che della Protezione civile con delega data alla Regione Veneto, Regione Veneto, ma anche la prefettura, i Vigili del fuoco, le Forze armate e tutto quello splendido volontariato che non conosce divisioni, né di parte, né di regioni, quando si tratta

che in questa circostanza ha voluto ricordare ancora una volta i fiumi di denaro che sono andati verso il Sud Italia senza alcuna utilità,

La Casa dei gladiatori rappresenta anche l'economia turistica di una Regione e bisogna aver rispetto, credo, anche di quella, come si ha rispetto ‑ e intendo averlo fino in fondo ‑ degli agricoltori, delle aziende,

nazionale. Lo dico da italiana del Mezzogiorno d'Italia.

semplicemente per esprimere - come già abbiamo fatto in modo informale ma accorato nei giorni scorsi - solidarietà alle popolazioni del Veneto e delle altre Regioni, colpite dalle avversità atmosferiche degli ultimi giorni, e per estendere questa solidarietà ai colleghi che le rappresentano dal punto di vista dell'espressione territoriale. Invece siamo costretti ad aggiungere a quei danni altri danni, a quei disagi altri disagi, a quella disperazione nuova disperazione.

nella Valle del Calore, nell'Alto Sele, nella Piana del Sele, in Penisola amalfitana (già, signor Sottosegretario, così tragicamente segnata dagli eventi del 9 settembre, in quella serata tragica che che comportò la scomparsa della giovanissima Francesca Manzi), nell'agro nocerino-sarnese, nella stessa città di Salerno, che è stata colpita anche lungo il litorale, con ingenti danni alla portualità turistica e alle imbarcazioni.

alle colture nelle zone che ho indicato, alle aziende zootecniche. Insomma, siamo di fronte ad una vera e propria calamità naturale. Davanti a questi fatti, sorge naturalmente spontaneo il solito proposito, che deve suonare però in quest'Aula come un impegno solenne da assumere da parte del Governo e delle forze politiche, anche contrapposte, ma unite di fronte a questa finalità: individuare l'antidoto, camminare sempre più lungo un percorso che guardi con attenzione alle attività di prevenzione. Lei sa bene, signor Sottosegretario, quanto la nostra provincia sia stata nel tempo drammaticamente segnata da eventi di natura idrogeologica per il noto dissesto che la affligge. Basti citare l'esempio di Sarno, di Siano e di Bracigliano, la tragica alluvione del 1998. Ella all'epoca non era nelle funzioni che poi avrebbe ricoperto, ma più recentemente ha seguito con attenzione - e le siamo grati anche per questo le tante opere che sono state poi costruite a difesa dell'abitato e naturalmente della pubblica incolumità. Semplicemente un messaggio conclusivo, che fa un po' eco a quello delle autorità istituzionali, a quello dello stesso presidente della Provincia di Salerno: la dichiarazione dello stato di emergenza per la Campania, per la provincia di Salerno in particolare, ma naturalmente un'esatta quantificazione del danno, e poi un fronte comune per mettere in campo iniziative adeguate sotto il profilo della prevenzione.

l'ha ridotta un acquitrino. I 500 millimetri di acqua che in poche ore hanno colpito il Veneto hanno provocato frane ovunque, una marea di fango che ha fagocitato ponti, strade, case, negozi ed aziende. Il bilancio catastrofico, ma non definitivo, purtroppo, è di più di 4.000 sfollati, 500.000 persone colpite; 131 sono i Comuni - l'ha detto anche lei - interessati dall'evento, con gravi danni agli argini dei fiumi, alle case e alle aziende.

che hanno perso tutto (casa azienda) e che caparbiamente cercano di salvare qualcosa tra le cose care che mestamente mettono fuori di casa e ammucchiano lungo le strade. Chi non ha visto non può immaginare l'ecatombe di piccole e medie imprese artigiane e agricole; la miriade di imprese artigiane e agricole appunto che con mutui e scadenze fiscali si ritrovano senza niente, con tutto sott'acqua, campi, animali e macchinari. Tutto andato; i sacrifici di un'intera vita ridotti in una poltiglia di fango ed acqua. Ma questa gente è là, con la Protezione civile, con i Vigili del fuoco, tanti volontari; è là perché vuole riprendersi al più presto la casa, i negozi e le proprie aziende, salvare il salvabile. La gente veneta non aspetta che altri facciano al loro posto, perché hanno l'orgoglio e l'abitudine di non stare con le mani in mano; prevale sullo sconforto e la disperazione la voglia del fare e fare presto. Ora la gente veneta ha chiesto aiuto. Il Veneto, che contribuisce con il 10,3 per cento del PIL nazionale, ha chiesto risorse per riprendere a vivere lavorando ed assicurare un futuro alla propria gente e ai suoi figli. Tutti capiscono che sarebbe un errore gravissimo, anche sotto il profilo economico per tutto il Paese, non far ripartire velocemente il motore produttivo veneto. Per questo motivo, tutti noi senatori del Veneto eravamo pronti a criticare i 20 miseri milioni stanziati per le cinque Regioni in emergenza. Ma dopo le promesse del nostro ministro Bossi durante la sua visita in Veneto, quando ha accompagnato il *premier* Berlusconi, la speranza si è riaccesa e, alla alla faccia dei parolai e dei contestatori, gli aiuti sono arrivati: 300 milioni di euro ed altri 450 sembra arriveranno dalla UE. Come veneto mi sento orgoglioso della mia gente, della forza che sta dimostrando. Con i sindaci in prima linea, mi sento di ringraziare tutti coloro che sono accorsi per dare aiuto e sostegno al popolo veneto: tutti i volontari, la Protezione civile, l'Esercito, i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Un grazie particolare al nostro presidente Luca Zaia che, con la sua pragmaticità, ha saputo essere vicino alla gente non con chiacchiere e passerelle TV, ma cercando fondi per la ricostruzione del nostro Veneto; fondi che sono arrivati. Un grazie a lei, dottor Bertolaso, per l'informativa e per il lavoro straordinario della Protezione civile da lei coordinata. Grazie infine a tutti i sottoscrittori dei contributi volontari destinati alla ricostruzione del Veneto. L'unica nota stonata è venuta dal ministro Galan - non ce l'aspettavamo - che ha detto: dai miei concittadini piagnistei eccessivi. Dopo una battuta del genere mi viene da pensare che forse, da quando si è trasferito a Roma, sta troppo chiuso nel Ministero ed ha perso il contatto con la realtà. Signora Presidente, cinque minuti per parlare della tragedia che ha colpito il Veneto sono un minutaggio un po' assurdo, e francamente non capisco con quali criteri venga organizzato il calendario dei lavori da parte dei Capigruppo. Spero che un minuto in più me lo concederà. Dobbiamo parlare di una tragedia che ha comportato tre morti ed ha colpito solo nel Veneto più di cento comuni, decine di migliaia di persone, centinaia di aziende. Devo però parlare anche dei gravi danni che si sono verificati in Liguria (a Genova e in altre città liguri), in Toscana, in Calabria e ora in Campania. Innanzitutto, esprimo la solidarietà del Gruppo del Partito Democratico alle famiglie dei deceduti e a tutti i cittadini che sono stati così duramente colpiti nei loro beni. Signor Sottosegretario, lei è stato nel Veneto ed ha potuto constatare personalmente la gravità dei danni per le famiglie e per le imprese, la loro estensione. Lei ha visto anche la straordinaria reazione della popolazione: ciò che hanno fatto i nostri sindaci, il personale comunale, i volontari della Protezione civile, le Forze armate, le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, gli operai delle aziende danneggiate gli organi dello Stato e della Regione. Li ringraziamo tutti, insieme a tanti cittadini italiani e stranieri che generosamente hanno aiutato le famiglie in difficoltà. Purtroppo, come lei ha osservato, migliaia di famiglie ancora non possono rientrare nelle loro case o vivono in case allagate, senza luce e riscaldamento, e moltissime imprese devono purtroppo ripartire da capo. non tutto è andato bene nel coordinamento territoriale, e mi dispiace dirlo. Troppi sindaci nelle prime ore hanno dovuto arrangiarsi da soli. Più tempestive allerte, specie nei comuni della bassa padovana, avrebbero consentito di limitare i danni, mettendo in salvo almeno una parte dei beni mobili. Hanno ceduto degli argini: non solo esondazioni, ma cedimento di argini. Non per caso, purtroppo: non possiamo dimenticare che negli ultimi cinque anni la Regione Veneto ha ridotto del 70 per cento il capitolo manutenzione e sistemazione di corsi d'acqua, e del 50 per cento i fondi per la sicurezza idraulica. Non meravigliamoci se poi ci sono delle conseguenze. Non possiamo dimenticare che per l'opposizione di alcuni sindaci della maggioranza politica nazionale non si sono realizzate casse di espansione, per le quali vi sono progetti esecutivi e finanziamenti già erogati, la cui realizzazione avrebbe consentito di limitare i danni. Non tutto è solo colpa della natura: vi è anche l'imprevidenza di chi governa. Ora lo Stato deve operare: è chiaro ciò che serve, non è purtroppo la prima calamità che ha effetti drammatici per i cittadini, e sarebbe ora, signor Sottosegretario, che lo Stato si dotasse di un sistema assicurativo che consenta di rendere certi gli interventi e la rifusione dei danni. Depositiamo in queste ore un disegno di legge contenente ciò che secondo noi va fatto: interventi a fondo perduto a favore delle famiglie e delle imprese daneggiate; sospensione degli adempimenti e dei termini di pagamento delle imposte statali e locali; sospensione degli studi di settore; detassazione degli investimenti finalizzati alla ripresa dell'attività produttiva; provvidenze di tutela sociale per chi resta senza lavoro. Le imprese devono avere la certezza che tutto ciò che serve per rimettersi in piedi subito sarà messo a disposizione. Per i Comuni, la sospensione del Patto di stabilità anche per le spese sostenute con fondi propri ed interventi straordinari di manutenzione delle opere pubbliche danneggiate. danneggiate. I Comuni siano i terminali degli interventi: no ad un nuovo centralismo regionale. Servono procedure rapide e semplici; servono fatti e non promesse, caro signor Sottosegretario, cari colleghi. Lei sa, signor Sottosegretario, che i cittadini colpiti da trombe d'aria che hanno interessato i comuni veneti negli ultimi due anni sono ancora in attesa di vedere soddisfatte le loro richieste nonostante le assicurazioni della Protezione civile a suo tempo formulate. Lei sa, signor Sottosegretario, che, per l'alluvione di Messina, dei 70 milioni promessi nulla è stato ancora erogato. Agisca perciò lo Stato, agisca l'Unione europea; bene se il Governo provvede ai primi stanziamenti di fondi, ma occorre che alle parole corrispondano fatti precisi, e i precedenti non sono del tutto confortanti. Saremo a fianco del Governo per ciò che di positivo verrà fatto e vigileremo perché alle promesse corrisponda il dovere dei fatti, subito, perché chi sta soffrendo non può aspettare e l'economia deve poter ripartire. Bisogna evitare che insieme all'acqua si ritiri l'attenzione dei *media* e delle istituzioni, perchè chi ha subito l'alluvione non può farcela da solo, e questo allo Stato deve essere chiaro.

a nome in modo particolare dei colleghi senatori veneti, qui autorevolmente rappresentati dal Ministro Sacconi che ringrazio subito,

quanto è accaduto, la relazione del Sottosegretario e questi primi interventi da parte del Governo. Desidero dire subito che chi pensò, nei giorni immediatamente successivi a questa calamità, di speculare politicamente su una vicenda che è solamente drammatica, triste...

provato a speculare su una vicenda tanto tragica, ha avuto una risposta oggi, la più pronta e la più autorevole, dopo la visita di ieri del presidente del Consiglio, Berlusconi,

sulla capacità di essere coerenti ed operativi rispetto alle circostanze purtroppo intervenute. Le cifre sono state ricordate dal sottosegretario Bertolaso, tutte: le risorse stanziate dal Governo, quelle che potranno arrivare dall'Unione europea, quelle messe a disposizione con interventi particolari da parte del sistema bancario; altre potranno essere trovate per venire incontro alle emergenze e anche agli investimenti che dovranno essere effettuati, in modo particolare dalla Regione, per mettere in maggiore sicurezza, per esempio, gli impianti idrovori

fondo la natura della nostra gente, come ricordava benissimo l'amico Cagnin prima di me. Voglio inoltre notare in modo particolare la presenza dello Stato, dello Stato, del troppo, a volte, deprecato Stato, nelle sue formazioni più autorevoli. Inizio dalla Protezione civile, carissimo sottosegretario Bertolaso, per passare alle forze dell'ordine, ai nostri Carabinieri, alla nostra Polizia di Stato, ai Vigili del fuoco, ai militari, alle organizzazioni tutte, statali e non statali, che hanno dimostrato che lo Stato c'è, che lo Stato esiste, che lo Stato è fatto da tutte le Regioni italiane, cara collega Poli Bortone, che lo Stato non intende minimamente far mancare il proprio aiuto alla gente del Veneto, che non che non è abituata a chiedere e quasi si vergogna chiedere, ma si è trovata in questa circostanza in condizioni realmente drammatiche. Quindi, grazie presidente Berlusconi; grazie Ministri veneti; grazie presidente della Regione, Zaia. Grazie, in particolare, carissimo sottosegretario, dottor Bertolaso,

in questi mesi, e il presidente Berlusconi, ieri, andando a Padova avete dimostrato, insieme, nel modo più bello, limpido ed autorevole, che non c'è amarezza che tenga rispetto alla soddisfazione alla grandezza che porta nel proprio intimo essere vicini alla propria gente con un servizio prezioso ed illuminato.

Ricordo che anche la Liguria, pure in modo più puntuale, ha avuto danni significativi. Finora gli stanziamenti sono di 10 milioni di euro; mi auguro che anche per la Liguria si possa trovare qualcosa in più, perché i danni sono davvero molto superiori.

al bando. Proprio in questi giorni nel Laos c'è una riunione internazionale di tutti i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Oslo. Tra questi Paesi c'è anche l'Italia: il nostro Paese ha sottoscritto questa convenzione, ma non l'ha ancora ratificata.

in considerazione dell'avanzato stato di attuazione dei procedimenti autorizzativi relativi al tratto Sulmona-Foligno e alla centrale di compressione di Sulmona.

La seduta è tolta Grazie